Onorevoli colleghi, come già comunicato per le vie brevi ai Gruppi parlamentari, poiché le Commissioni di merito non hanno ancora concluso l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge all'ordine del giorno, la seduta inizierà con l'esame del successivo punto all'ordine del giorno del Governo, colleghi senatori, la relazione della Commissione straordinaria per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati sull'attività svolta negli anni 2009 e 2010

I nostri lavori hanno preso il via da una mozione, anch'essa a firma di tutti i Capigruppo, approvata nell'ottobre 2008.

effettivamente di crisi, nel quale si assisteva al più ampio e veloce aumento dei prezzi a partire dagli anni Settanta. Il prezzo del petrolio era aumentato

L'aumento dei generi alimentari aveva seguito di poco quello del petrolio, e gli incrementi percentuali maggiori riguardavano proprio il costo dei cereali e dell'olio commestibile. Da cosa è dipeso il tutto? Era innegabile che l'aumento esponenziale del costo del petrolio fosse legato in parte preponderante anche a comportamenti speculativi. Infatti, l'incremento patologico del prezzo dei prodotti petroliferi testimonia che la presenza di comportamenti speculativi favoriti da numerosi passaggi commerciali, che iniziano con l'estrazione del greggio e terminano con l'utilizzazione del carburante. Il problema del contrasto del fenomeno inflattivo e del controllo dell'incremento del prezzo al barile del petrolio assumeva allora un rilievo centrale, oltre ad assumerlo anche oggi in tutto l'ambito internazionale.

sottolineando che i rincari delle materie prime ponevano una minaccia alla crescita dell'economia globale, ma non individuava alla fine alcun piano di azione per contrastare tutte le turbolenze dei mercati sui prodotti petroliferi. Sempre quel G8 soffermava l'attenzione sull'esigenza di effettuare uno studio dei fattori reali e finanziari alla base del rialzo dei prezzi del petrolio e delle materie prime e affidava a tale scopo l'incarico al Fondo monetario internazionale e all'Agenzia internazionale per l'energia. La stessa Commissione europea affrontò, sempre nello stesso anno, questo problema nel tentativo di formulare risposte adeguate ad attenuare gli effetti dell'aumento mondiale dei prezzi, e specificatamente di quello dei combustibili; dei combustibili; propose inoltre misure per la promozione dell'efficienza energetica a livello aziendale nonché familiare. La stessa Commissione invitò allora tutti gli Stati membri a prendere iniziative a breve termine per sostenere le fasce più povere della popolazione.

raggiunta nel mese di giugno - arrivando ai massimi livelli dal 1996. I beni che registravano il maggiore incremento risultavano quelli alimentari e i carburanti. In questo contesto, a soffrire particolarmente del rialzo dei prezzi dei prezzi sono le famiglie, soprattutto quelle a basso reddito e a reddito fisso, le quali rischiano di vedere compromesso il potere di acquisto, con effetti negativi anche sul ciclo economico per l'indebolimento della domanda interna. Le azioni che sono state messe in atto dal Governo iniziarono con la finanziaria per il 2008, la quale ha introdotto una nuova disciplina in materia di sorveglianza dei prezzi e ha attribuito a ciascuna camera di commercio il compito di rendere noto al pubblico

presso il Ministero dello sviluppo economico, che corrisponde al Garante per la sorveglianza dei prezzi. Successivamente, con il decreto-legge n. 112 del 2008, si sono ulteriormente ridefinite le funzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi, attribuendo a tale figura il compito di analizzare le segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento, nonché la possibilità di convocare imprese ed associazioni di categoria al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo.

che affrontando a livello nazionale e internazionale le tematiche di cui in premessa. A tale scopo, infatti, è stata deliberata l'istituzione della Commissione straordinaria per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati, mozione approvata all'unanimità il 7 ottobre 2008.

Le audizioni messe in atto ci hanno consentito di individuare le principali cause delle speculazioni sui prezzi del mercato economico italiano. Secondo i dati emersi, l'inflazione italiana è sostanzialmente allineata alle rilevazioni della media dell'eurozona. Nel biennio 2007-2008, nonostante il rallentamento dell'economia mondiale e la successiva recessione, si è registrato un rapido aumento dell'inflazione in tutta l'eurozona. In Italia l'inflazione ha registrato in questi ultimi anni un'accelerazione, provocata in prevalenza dalle componenti alimentare e energetica, che incidono sull'indice generale dei prezzi al consumo per una percentuale di circa il 25 Nel 2009 si è rilevata una discesa dell'inflazione a livello internazionale, per lo più dovuta al prolungarsi degli effetti della crisi. prezzi dei prodotti industriali ha iniziato a rallentare nel dicembre 2008 fino al gennaio 2010. Nel 2009 i prezzi alla produzione del manifatturiero sono scesi del 4,8 per cento; nello stesso anno, tessile e abbigliamento sono cresciuti meno dell'inflazione. Il dato tendenziale della discesa dei prezzi della produzione generale 2010 è pari a meno 0,8 A gennaio 2010 i prezzi dei prodotti industriali del settore manifatturiero sono saliti dello 0,7 per cento. L'unico comparto ad essere cresciuto notevolmente più dell'inflazione è il settore dei prodotti petroliferi (ed è per quello che ci siamo concentrati particolarmente su questo ambito),

In generale si è rilevato che i bassi livelli di inflazione, almeno fino al primo semestre 2009, sono stati causati per lo più dalla riduzione dei prezzi energetici. La deflazione dei prezzi alla produzione industriale, per molti comparti, in Italia è stata più intensa rispetto all'area euro. Anche in un comparto protetto dalla concorrenza come quello dei servizi pubblici locali non energetici (acqua, raccolta rifiuti, trasporto pubblico eccetera) i prezzi in Italia negli ultimi cinque anni sono cresciuti del 33,1 per cento, contro il 16,6 della media dell'eurozona. La necessità di comprendere le dinamiche della crescita dei prezzi e il conseguente impoverimento progressivo dei consumatori hanno indirizzato pertanto il cammino della Commissione verso l'acquisizione di informazioni, elaborazioni e proposte volte al contenimento delle manovre speculative e degli effetti dell'inflazione. Passiamo alle audizioni. Secondo l'ISTAT, quando l'inflazione accelera l'aumento dei prezzi è maggiore in Italia rispetto alla media dell'eurozona (si amplia la nostra spinta inflazionistica); quando invece il tasso di crescita dei prezzi inizia a scendere si rileva che scende meno velocemente in Italia che nella media europea: ciò dipende non solo dagli impulsi esogeni, ad esempio dall'aumento del prezzo del petrolio, ma anche dall'inflazione fatta in casa, quella che decelera meno rapidamente. Unioncamere segue questo quadro: alla fine del 2008 l'indice dei prezzi armonizzati (che è quello usato per confrontare i Paesi dell'area euro) segna un aumento del 2,4 per cento in Italia, rispetto all'1,6 della media europea. Ciò è dovuto soprattutto ai ritardi con cui si trasmettono sia nella filiera dell'energia sia, ancor di più, in molte filiere alimentari, le inversioni dei prezzi internazionali.

Si sommano così potere di mercato e inefficienze. Unioncamere sottolinea la frammentazione e sovrapposizione di competenze tra Stato, Regioni e Province sul settore. Inoltre ricorda l'importanza di un'azione volta a diffondere la conoscenza precisa ed articolata sui prezzi e sulle condizioni dell'offerta. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato in audizione ha evidenziato che essa stessa è chiamata frequentemente ad aprire procedimenti nei confronti di operatori del settore del credito al consumo con riferimento ai messaggi pubblicitari diffusi per la non veridicità degli stessi o la difficoltà di individuare le condizioni di erogazione dei finanziamenti. La rilevanza della forte variazione del prezzo del petrolio e della successiva trasmissione al prezzo al consumo sono analizzate nella relazione dell'Autorità. Sono emersi i molti limiti della struttura distributiva: troppi impianti, di piccola dimensione, senza altri prodotti, con troppa manodopera. Nell'audizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas è stata analizzata la misura e la qualità della competizione nel processo di liberalizzazione che ha caratterizzato gli ultimi dieci anni nella filiera dell'energia.

60 per cento delle famiglie italiane) ha pagato l'elettricità meno dell'80 per cento della media europea. Le altre famiglie, con consumi maggiori o per le seconde case, hanno invece pagato l'energia più della media europea. Le imprese italiane hanno pagato per l'elettricità prezzi più elevati della media europea, a volte anche del 35 per cento. Le bollette del gas per le famiglie italiane sono state inferiori a quelle medie europee per le famiglie che usano il gas solo per consumi contenuti. Gli altri consumi sono stati in linea con la media europea. I prezzi per il gas pagati invece dalle imprese, in particolare per le classi di consumo basse e intermedie, sono stati su livelli molto vicini alla media europea. alla media europea. Dopo la Danimarca, l'Italia è il Paese con le imposizioni sul chilowattora per utenze non domestiche, al netto dell'IVA, più alte d'Europa. Per il mercato del gas è difficile parlare di concorrenza. I concorrenti del principale distributore nazionale non arrivano al 10 per cento del mercato all'ingrosso. Per questo motivo non si sviluppa il mercato al dettaglio. L'operatore dominante ENEL è sempre in grado di «fare il prezzo» e di imporlo, per ricavare extraprofitti anche nei momenti di discesa dei prezzi. Dall'audizione della Banca d'Italia possiamo dedurre che in Italia la riduzione dei tassi d'interesse, seguita alla riduzione dei tassi ufficiali della BCE dopo l'ottobre 2008, è allineata con i valori registrati nella media dell'area dell'euro. Anche per le famiglie italiane la situazione appare di recente migliorata (pensiamo al decreto del ministro Tremonti per la rinegoziazione dei mutui). In passato, infatti, la rinegoziazione dei prestiti contratti era più onerosa in Italia rispetto alle famiglie degli altri Paesi dell'area dell'euro. La Banca d'Italia osserva l'eccessiva proliferazione della gamma degli strumenti bancari proposti alla clientela: tipico è il caso dei conti correnti. Di fatto questo ostacola la necessaria comparazione ed una scelta più avveduta e più consona ai propri interessi. Le ricerche svolte in materia, illustrate dalla Banca d'Italia ed operate dall'Autorità garante della concorrenza e del e del mercato, hanno dimostrato che i costi di un conto corrente sono maggiori in Italia rispetto a quelli rilevati negli altri principali Paesi europei. È necessaria pertanto un'azione per aumentare l'effettiva trasparenza e la comparabilità delle condizioni offerte dalle diverse banche. Giunge a proposito l'opportunità che abbiamo oggi, in sede di 14ª Commissione, con riferimento alle osservazioni in fase ascendente della proposta di direttiva del Parlamento europeo al Consiglio in al Consiglio in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali, di trasferire il lavoro operato in Commissione sotto forma di parere al Parlamento europeo. europeo. Nella proposta che ci accingiamo a sottoporre alla 14ª Commissione chiederemo al riguardo un'integrazione con pochi dati, dicendo che sembra opportuno che venga prevista la predisposizione di contratti standard aventi un contenuto omogeneo, sintetico, facilmente intelligibile. In tal modo i consumatori possono comparare le condizioni richieste dai vari istituti eroganti il credito e scegliere in maniera informata il prodotto che meglio soddisfa le proprie esigenze. Si è rilevata una ripresa dei prestiti e dei finanziamenti alle famiglie ed alle imprese nel secondo semestre 2010, ancora condizionati dal deterioramento della qualità del credito per la passata recessione. I tassi degli interessi bancari sui prestiti alle famiglie e anche alle imprese sono diminuiti in tutta l'area euro, con la sola eccezione per i tassi sul credito al consumo. Nel 2010 Bankitalia ha utilizzato i propri poteri ispettivi e di indagine per sanzionare violazioni sulle informazioni ai consumatori. È stata infatti imposta una maggior trasparenza agli operatori sulle condizioni praticate alla clientela. Parzialmente diverse invece sembrano le posizioni dell'Associazione bancaria italiana, ABI. Infatti, secondo ABI, i servizi finanziari non hanno contribuito alla crescita dell'inflazione, ma hanno anzi favorito una sua attenuazione.

in Italia si è osservata una dinamica generalmente più contenuta dei prezzi dei servizi finanziari. Interessanti sono stati gli spunti che ci ha offerto l'audizione della Guardia di finanza, la quale compie, lo ricordo, costanti attività di monitoraggio generale dei prezzi al consumo. Vengono svolte attività di indagine conoscitiva, su richiesta del Garante per la sorveglianza dei prezzi. Sono emerse interessanti considerazioni in merito al credito al consumo. I prodotti di credito al consumo vengono proposti dalle banche tramite società finanziarie, promotori, agenti e così via. I messaggi pubblicitari di tali prodotti sono stati spesso sanzionati perché omissivi sui prezzi reali dei prodotti proposti. Anche sui mutui, alcuni accertamenti della Guardia di finanza hanno accertato che mediante il prestito immobiliare fino a quasi tutto il 2008 le persone non solo pagavano il prezzo della casa, ma anche le provvigioni all'agente immobiliare, gli onorari e le imposte dovute al notaio. al notaio. Si è arrivati a concedere prestiti fino al 53 per cento del reddito disponibile nel rapporto tra rata e debito. I mutui sono stati concessi principalmente nella forma del prestito indicizzato al costo del denaro o suoi derivati (ad esempio l'Euribor). Il rapporto tra rata e reddito era già poco sostenibile allora, con i mutui indicizzati ad un costo del denaro che variava attorno all'1,5 per cento. Quando il costo del denaro è salito di circa quattro punti, tutto il meccanismo è saltato, e le ripercussioni sul mercato immobiliare le abbiamo potute notare tutti. Un altro tema affrontato è quello delle carte *revolving*. Sono carte che mettono a disposizione dell'utente una vera e propria riserva di denaro sulla quale contare per effettuare acquisti o prelievi di contante. Il cliente si impegna a restituire gli importi utilizzati rispettando un importo di rata minima mensile stabilita precedentemente in contratto. Gli interessi sulle carte *revolving* dovrebbero essere calcolati in base a due parametri: il TAN (tasso annuo nominale ) e il TAEG (tasso annuo effettivo globale, che tiene conto di tutte le spese L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti di una delle più importanti società di carte di credito e di altre otto banche e società finanziarie, per possibili intese restrittive della concorrenza e poca chiarezza espositiva dei prodotti.

Si stima che, tra rimborso di capitale, interessi, mascherate commissioni di istruttoria e mediazione, si arrivi anche al 30 per cento del capitale preso a prestito. In una denuncia si è rilevato un tasso d'interesse del 54,21 per cento, notevolmente superiore alla soglia di usura. La Guardia di finanza ha proceduto ad ispezioni, e in tre casi limite è emerso che ad alcuni soggetti sono stati applicati tassi del 46,32, del 108,99 e del A mettere in allerta circa i rischi di insolvenza relativi a questo utilizzo delle carte di credito è stato anche un rapporto del 2009 del Fondo monetario internazionale. alcuni settori economici, e in particolare a quello dei panificatori e dei produttori di pasta, su richiesta del Garante, la Guardia di finanza ha compiuto alcuni accertamenti. I panificatori di certe zone italiane sono stati scoperti nel concordare

ha negato posizioni di cartello tra i produttori. I rincari registrati nel prezzo al consumo non sono stati della stessa incidenza della materia prima. Secondo l'Associazione italiana panificatori il costo della materia prima incide solo per il 12 per cento sul costo finale del pane, aumento è dovuto principalmente al forte incremento della produzione di biocarburanti a scapito della coltivazione del grano e alle fasi di intermediazione della filiera. Simili gli accordi sui prezzi trovati dalla Guardia di finanza nel commercio al dettaglio del burro nelle province di Palermo e Reggio Calabria e sul prezzo del latte per l'infanzia a Roma, Milano, Napoli e Palermo. Sempre un accordo di cartello è stato provato nelle indagini sulla filiera cerealicola. Al consistente decremento del prezzo del grano sui mercati internazionali non è corrisposta una flessione dei prezzi delle farine e della semola. Il risultato per la pasta, come prodotto derivato, è stato che non ha avuto

L'Unione industriali pastai non ha negato il cartello sui prezzi accertato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, però sostiene che delle 28 imprese coinvolte 16 hanno chiuso i bilanci in rosso:

animale è stata provata un'intesa restrittiva della concorrenza che ha procurato danni al mercato italiano e comunitario. Sono state controllate 267 filiere distributive di cinque prodotti ortofrutticoli (cavolfiore, lattuga romana, zucchine di serra, arance tarocco e mele golden):

Dall'audizione di Confesercenti è emerso che gli incrementi del prezzo dei beni alimentari sono dovuti sostanzialmente a variabili esogene e speculative esterne al settore distributivo. Ad esempio, viene citato il prezzo della farina e dei suoi derivati. L'aumento delle tariffe sui rifiuti solidi urbani e sull'acqua di oltre il 40 per cento in questi ultimi anni ha indubbiamente aggravato in modo significativo i costi per gli esercenti. Secondo Confindustria, il divario sui prezzi al consumo tra l'Italia e Nazioni europee come la Germania provocherà un'erosione di competitività, con ripercussioni sulla crescita e sull'occupazione. La maggiore inflazione riduce il potere d'acquisto delle famiglie e produrrà sicuramente una riduzione del valore reale delle retribuzioni. È aumentato il divario tra Italia ed Europa sull'inflazione *core*, e questo è dovuto ai prezzi dei servizi praticati in Italia. I prezzi al consumo dei beni industriali non alimentari e non energetici, secondo Confindustria, sono stati la componente più misurata dell'inflazione italiana. L'aumento dei prezzi al consumo ha diminuito il potere di acquisto delle famiglie, quindi i consumi, cosa che sta penalizzando la redditività e anche gli investimenti delle imprese. imprese. In conclusione, purtroppo le condotte anticoncorrenziali ai danni dei consumatori rimangono, nel nostro Paese, non sanzionabili dal punto di vista penale e amministrativo, fino a quando non influiscono sull'intero mercato nazionale. Vengono analizzate e scoperte anomalie che contrastano con gli equilibri tra domanda ed offerta nel mercato. Tutto però rimane senza conseguenze, salvo che le condotte poste in essere non configurino limiti alla concorrenza di mercato, ossia cartelli illegali per condizionare i prezzi dei beni venduti. Come evidenziato nella relazione della Guardia di finanza, bisognerebbe adeguare le previsioni di legge alla gravità dei fenomeni di manipolazione dei prezzi. Le due principali fattispecie di reato previste dal codice penale in materia di prezzi, l'articolo 501 (aggiotaggio) e il 501*-bis* (manovre speculative su merci), risultano complesse e di difficile applicabilità; si lasciano impunite pertanto singole violazioni che non incidano sull'intera collettività. Uno dei settori che più riverbera gli aumenti di prezzo su tutti gli altri beni è il settore degli energetici. Il controllo stretto delle tariffe di elettricità e gas è garantito dall'Autorità dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che annovera fra i suoi fini specifici proprio la definizione di sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti. Per quanto riguarda i carburanti, invece, si è potuto notare come si tratti di un settore del tutto anomalo. Il prezzo del greggio è infatti controllato da pochi produttori che ne fissano il prezzo indipendentemente dalla domanda e dall'offerta del momento. A tale anomalia se ne aggiunge un'altra: la stessa compagnia che gestisce estrazione, trasporto, raffinazione, distribuzione e vendita al dettaglio non garantisce chiaramente un livello di concorrenza e di competizione sul mercato. Una filiera così rigida pertanto, in cui si realizza una scarsa concorrenza, non produce effetti positivi sui prezzi finali del prodotto. Per ovviare a ciò sono stati presentati da componenti la Commissione i disegni di legge n. 2636) in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, tesi a rendere più autonoma la figura del gestore dell'impianto, e in grado di approvvigionarsi sul mercato ponendo ponendo in concorrenza le varie compagnie e realizzando così sensibili risparmi per gli acquirenti finali. Infine, la Commissione ha preso atto che in numerosi contesti la presenza di asimmetrie informative, la mancanza di

da pratiche che comprimono l'imprenditorialità dei gestori e puniscono i consumatori (è il caso della distribuzione dei carburanti) e, sopratutto, lo scarso affermarsi della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas, determinano la necessità che Parlamento e Governo assumano le indispensabili iniziative per favorire il migliore dispiegarsi del mercato e le liberalizzazioni necessarie a stimolare la concorrenza, nonché le misure atte a tutelare i contraenti deboli quali i consumatori, soprattutto quelle fasce più anziane e meno informate della popolazione. In tal senso, la Commissione invita anche il Governo ad esercitare la delega prevista nella legge n. 99 del 2009 e a presentare il disegno di legge annuale per la concorrenza, non ancora approdato in sede parlamentare. Il documento che ho illustrato è stato approvato all'unanimità dalla Commissione il 29 marzo. Devo ringraziare tutti i colleghi per la collaborazione data nonché per i contributi fattivi alla stesura di questa relazione.

di cui la Commissione si avvale: il professor Giacomo Vaciago, ordinario di politica economica presso l'università «Cattolica» di Milano e direttore del LAM, Laboratorio di analisi monetaria; l'avvocato Agostino D'Antuoni, presidente di «Avvocati per le riforme» nonché presidente del Centro studi parlamentari; il giornalista economico dottor Simone Baiocchi. Ringrazio questi consulenti tecnici per le competenze professionali che ci hanno offerto,

Quello che si evidenzia è che nel nostro Paese l'andamento dei prezzi produce tendenzialmente un effetto inflattivo maggiore rispetto al resto della zona euro.

abbastanza stabilito che accelera quando la spinta inflazionistica europea è maggiore e decresce con maggiore lentezza quando decresce quella europea. Abbiamo cioè un andamento abbastanza asincrono rispetto alla situazione dell'eurozona, e ciò dipende non soltanto da impulsi esterni al nostro sistema,

L'inflazione è da anni sopra la media nazionale nel Mezzogiorno e nelle isole e vi è una vischiosità nel rientro che caratterizza soprattutto i prezzi alimentari e quelli energetici. Le ragioni della minore reattività delle dinamiche dei prezzi nel nostro Paese sono legate a un peggiore funzionamento dei mercati, alla totale o parziale mancanza di concorrenza in numerosi settori, alla totale o parziale mancanza di trasparenza (come dicono le conclusioni), alla opacità e all'incomprensibilità delle offerte in altri settori, alla inefficienza delle reti distributive e al perdurare di forti asimmetrie informative. Sostanzialmente l'economia italiana, attraverso questa visione di insieme che la Commissione prezzi produce, ci racconta che in numerosi settori il problema è il funzionamento competitivo dei mercati interni. È piuttosto rivelatorio, a questo proposito, l'andamento dei servizi pubblici. Le tariffe dei servizi pubblici regolamentati sono quelle che crescono di più, mentre i servizi in concorrenza (cioè quelli non regolamentati) hanno una tendenza minore alla crescita.

a recuperare i costi sempre a spese del consumatore e non dell'efficienza produttiva. Per questo, nella parte conclusiva della relazione

che impegna il Governo a presentare il disegno di legge annuale per la concorrenza. La delega che il Parlamento ha votato con la legge n. 99 nel 47 «disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori».

in Italia vi è un maggiore incremento dei prezzi dei servizi e dei beni industriali non energetici. Nel 2010 si è registrato un maggior incremento dei prezzi al consumo degli energetici non regolamentati rispetto a quelli regolamentati, ma i servizi regolamentati crescono di più di quelli non regolamentati.

nell'offerta bancaria, cioè nei servizi che le banche offrono alla propria clientela. La Banca d'Italia mette in evidenza un *surplus* di offerta di modalità di accesso al conto corrente nelle banche italiane, peraltro fatta spesso con modalità del tutto fantasiose, sempre a discapito della trasparenza, della possibilità di valutazione da parte del cliente, del consumatore che si trova totalmente in balia dell'offerta predisposta. La Banca d'Italia segnala inoltre, assieme alla Guardia di finanza, come questa opacità di offerta abbia determinato una dinamica dei costi dei conti correnti per il consumatore normale più elevata di quella degli altri Paesi europei; inoltre, i servizi bancari sono in generale più elevati rispetto a quelli degli altri Paesi europei quando poi non si entra, sempre per l'opacità dei mercati

Numerosi prodotti, soprattutto legati al credito al consumo, hanno tassi di interesse enormemente più elevati del tasso di usura;

un costo per l'utenza non evidenziato negli accordi iniziali. Tutto ciò produce un maggior indebitamento delle famiglie,

l'oggetto di competenza del mutuo stesso; vi è un indebitamento che non è nelle previsioni di una singola famiglia, proprio per l'abuso di opacità.

le alterazioni della concorrenza e le ricadute sulla clientela avvengono principalmente a livello territoriale e in singoli mercati locali. Questo non fa scattare l'intervento dell'Autorità garante della concorrenza, se questa non viene messa in condizione, magari attraverso le camere di commercio, di operare anche sul controllo territoriale delle dinamiche domanda-offerta. In ultima analisi, di questo documento, oltre al resoconto che è stato fatto, è particolarmente importante la richiesta pressante fatta al Governo

e, contemporaneamente, affinché si agisca con maggiore rigore in tutte quelle forme di distorsione della concorrenza, di abuso della posizione dominante, di asimmetria informativa nei confronti del consumatore perché in settori delicatissimi (dal settore dell'energia a quello assicurativo, dal settore bancario alla filiera alimentare, e così via) la disorganizzazione sul versante dell'offerta e logiche di cartello o accordi sottobanco di natura monopolistica tendono ad alterare il mercato mercato e a far pesare l'eccessivo costo della disfunzionalità del mercato stesso sulle famiglie e sul consumatore più debole. Il messaggio che viene dalla Commissione prezzi è finalizzato ad una maggiore efficienza da parte di tutte le autorità, e in particolare dell'autorità di Governo, nel predisporre quelle normative che consentano al mercato di funzionare al meglio, correggendo le distorsioni che il mercato italiano presenta rispetto ai mercati europei.

che avrebbero il dovere di controllare sulle anomalie di prezzi e tariffe

fa, non avendo probabilmente gli strumenti per difendersi dalle accuse dei consumatori circa una speculazione sul cambio lira-euro, inventò addirittura l'inflazione percepita, per cui le famiglie hanno pagato un durissimo prezzo anche al cambio del segno monetario. Questo è un Paese dove

condizionano l'operato del Governo e della maggioranza. Lo abbiamo visto. Il minimo di tutela per un mercato che si dichiara libero riguarda la tutela che bisogna offrire ai consumatori per difendersi dai monopoli e dai cartelli attraverso la cosiddetta azione di classe. Ebbene, l'azione di classe, realizzata con grande fatica e che offriva la possibilità a tanti risparmiatori truffati

vuole, insieme alla CONSOB del presidente Vegas si inventano i *bond* da banco per indurre le famiglie a sottoscriverli e quindi risolvere i problemi

soprattutto alcuni Governi si inginocchiano di fronte ad un agire economico che deve essere lasciato a briglia sciolta e che è allergico alle regole. L'*Antitrust*, una delle poche autorità che fa il suo mestiere, sembra sia vissuta come un intralcio all'agire economico. Le relazioni che invia al Parlamento sono disattese e addirittura le si tagliano personale

le banche inventano nuovi balzelli e ogni giorno mettono le mani nelle tasche dei cittadini, non solo con i tre euro per prelevare contante allo sportello. Ci rendiamo conto?

e che possono detrarre nella dichiarazione gli interessi passivi. È un diritto del mutuatario avere la certificazione di quali tassi di interesse ha pagato, per poterli detrarre in sede di dichiarazione dei redditi: sapete quanto costa la certificazione,

dobbiamo affrancarci dal sistema bancario. Noi il primo atto lo abbiamo compiuto quando abbiamo approvato il milleproroghe. Ci sono cittadini che con grande fatica vanno in tribunale, impiegano decenni per far affermare i propri diritti contro i soprusi e gli abusi bancari, ottengono sentenze ripetute da parte della Cassazione, anche a sezioni unite, su quella pratica illegale denominata anatocismo (degli interessi sugli interessi) e poi arriva, come primo atto, il Governo e cancella tutto. Adesso abbiamo dovuto scomodare la Corte costituzionale, che si dovrà pronunciare per una norma che sicuramente è incostituzionale. Poi, il secondo atto è nello sviluppo: ma qual è lo sviluppo? È quello dei banchieri? Quello che si spaccia per aiuto alle famiglie che hanno i mutui intaccando la legge n. 108 del 1996, la legge antiusura?

per cento. Quindi il Ministro dell'economia comincia a fare politica monetaria, togliendo magari il lavoro alla Banca centrale europea, aumentando i tassi soglia del 79,9 per i tassi variabili, del 43

e non si fa nulla, anzi si assecondano i *desiderata* degli assicuratori, che vengono in Parlamento e si fanno approvare leggi contro i diritti dei consumatori e degli assicurati: in alcune zone,

ci sono le Autorità che dovrebbero fare le Autorità, come l'ISVAP, la CONSOB, la Banca d'Italia. Abbiamo grandi gruppi, grandi compagnie di assicurazione, come Fondiaria-SAI,

quindi, si dà anche una interpretazione amicale su quelle che sono le norme. Incidentalmente, a proposito della famiglia Ligresti indebitata con le banche,

noi. Caro presidente Divina, cari colleghi, se vogliamo che questo Paese esca dalle secche non dobbiamo guardare in faccia nessuno. Quando questi signori lobbisti si presentano Parlamento ad imporre norme che vanno contro i diritti dei consumatori, diamo loro il benservito. Solo in questo modo faremo ripartire il Paese.

La relazione che ci ha presentato contiene quindi molte informazioni puntuali. Esse ci restituiscono però un'immagine che, in fondo, nelle sue linee essenziali, conoscevamo già. La relazione apre con una descrizione dell'andamento

proprio in riferimento agli altri indicatori fondamentali dell'economia - il tasso di crescita, la disoccupazione, i conti con l'estero e (aggiungo io, perché la relazione non lo fa) lo stato della finanza pubblica

da un eccessivo o troppo rapido tasso di crescita, e non è il nostro caso), nella sostanza non possiamo definirci in linea con l'eurozona. Le informazioni derivanti dalle audizioni e dalle statistiche riportate nella relazione vanno ricondotte

nei tempi recenti, è molto rilevante lo *shock* della crisi internazionale, cui facevo riferimento prima. L'inflazione, quindi, si presenta fondamentalmente di due tipi: quella da domanda, dovuta ad una crescita troppo veloce, rispetto alla quale l'offerta non si adegua nei tempi giusti e, quindi, ne risente il sistema generale dei prezzi; e l'inflazione da offerta o da costi, laddove ci sono degli elementi del sistema produttivo che producono sistematicamente o strutturalmente a costi superiori alla media perché in questi elementi del sistema produttivo ci sono problemi non risolti. Da noi, purtroppo, l'inflazione è soprattutto da costi, a parte una componente rilevante dell'inflazione da domanda, cioè quella finanziaria derivante dallo stato dei nostri conti pubblici, purtroppo assai peggiore rispetto a quella degli altri Paesi con cui ci confrontiamo. ma sistematica, e strutturalmente fuori dagli standard e dalle medie dei nostri *input*, suggerisce che i risultati di questa relazione non sono da prendere sottogamba e devono invece indurci ad azioni più forti

argomento, ma purtroppo rimane uno dei nodi non risolti nel funzionamento dell'economia italiana. Si accumulano rendite, non esistono regole e sanzioni, si formano cartelli, e via È evidente che, essendo questi settori molto trasversali, ciò tende a trasmettersi a tutti i settori dell'economia che acquistano beni o servizi dai trasporti, dall'energia e dal credito. Di conseguenza, l'inflazione da costi si trasmette all'intero sistema economico.

È una inflazione principalmente da costi, e questo è più grave di quanto si pensi, perché, in situazioni di scarsa o peggiore crescita economica, che è esattamente la situazione che stiamo attualmente vivendo, l'inflazione va avanti per i fatti suoi e può facilmente farci scivolare nel pericolo della stagflazione, ossia dell'inflazione senza crescita, che più o meno abbiamo già ma che potrebbe anche peggiorare. Naturalmente da questo discende l'esigenza di misure strutturali che riguardano ‑ è evidente ‑ la concorrenza dei mercati e quindi le liberalizzazioni, la creazione di quelle norme e la predisposizione di quei controlli che la relazione stessa riconosce mancare. Vorrei però aggiungere che nel nostro Paese serve una cultura del mercato più che dei controlli. Probabilmente nel breve periodo abbiamo bisogno di maggiori controlli, ma nel lungo periodo dobbiamo renderci conto che i mercati devono funzionare

È un campanello d'allarme. Se non ce ne siamo occupati in quella occasione, dovremmo occuparcene molto presto, a cominciare dalla legge sulla concorrenza e naturalmente, negli anni a venire, nel Programma nazionale di riforma.

purtroppo le condotte anticoncorrenziali ai danni dei consumatori rimangono, nel nostro Paese, non sanzionabili dal punto di vista penale e amministrativo, fino a quando non influiscono sull'intero mercato nazionale. Nell'audizione del rappresentante della Guardia di finanza è emersa chiaramente la mancanza di strumenti di contrasto e di deterrenza alla crescita anomala dei prezzi. Vengono analizzate e scoperte anomalie che contrastano con gli equilibri tra domanda e offerta nel mercato. Ma tutto questo rimane senza conseguenze, salvo che le condotte poste in essere non configurino limiti alla concorrenza di mercato, ossia cartelli illegali per condizionare i prezzi dei beni venduti. L'allungamento della filiera con la presenza di molti intermediari tende ad incrementare i margini degli intermediari, producendo consistenti aumenti dei prezzi per il consumatore finale. Dal punto di vista normativo, come evidenzia la relazione della Guardia di finanza, bisognerebbe adeguare le previsioni di legge alla gravità dei fenomeni di manipolazione dei prezzi, ma le due principali fattispecie di reato previste dal codice penale in materia di prezzi, all'articolo 501 (aggiotaggio) e (manovre speculative su merci), risultano complesse e difficilmente applicabili. Sono infatti considerati da queste norme solo eventi di grandi dimensioni e si lasciano impunite le singole violazioni che non incidono sull'intera collettività. Spesso le manovre speculative sui prezzi hanno una rilevanza locale, come le comunicazioni fraudolente rivolte a gruppi di privati acquirenti. In assenza di norme precise per la violazione delle dinamiche di libero mercato vengono compiuti atti destinati a rimanere impuniti. Non viene colto il pericolo che alterazioni della normale crescita dei prezzi possono portare all'ordine pubblico e alla sicurezza economica. L'alterazione dei prezzi determina violazioni degli equilibri di concorrenza nelle produzioni industriali. I macroimpulsi inflattivi che si trasmettono sui prezzi per dinamiche globali sono aggravati dalle libere speculazioni spesso non sanzionabili. Uno dei settori che più riverbera gli aumenti di prezzo su tutti gli altri beni e servizi è il settore degli energetici. Il controllo stretto delle tariffe di elettricità e gas è garantito dall'*Authority* a ciò predisposta, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che annovera fra i suoi fini specifici proprio la definizione di sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti. Invece, per quanto riguarda i carburanti, si è potuto notare come si tratti di un settore del tutto anomalo. Il prezzo del greggio è controllato dai pochi produttori e fissato indipendentemente dalla domanda e dall'offerta del momento. A tale anomalia se ne aggiunge poi un'altra: talvolta la stessa compagnia gestisce estrazione, trasporto, raffinazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei combustibili; una filiera rigida, in cui si realizza una concorrenza per forza di cose scarsa, che sicuramente non produce effetti positivi sul prezzo finale dei prodotti. Per ovviare a ciò - rileva la Commissione nella sua relazione finale - sono stati presentati alcuni disegni di legge (Atto Senato n. 2283 e Atto Senato n. 2636) in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, tesi a rendere più autonoma la figura del gestore dell'impianto, e in grado di approvvigionarsi sul mercato ponendo in concorrenza le varie compagnie, realizzando così sensibili risparmi per l'acquirente finale. La Commissione ha preso atto che molto spesso la dinamica dei prezzi, oltre che essere il risultato dell'equilibrio sempre variabile tra domanda e offerta, è in numerosi settori sottoposta a fenomeni di alterazione della concorrenza, di costituzione di cartelli in grado di alterare il mercato, di pesanti e irragionevoli reti distributive sul versante dell'offerta, con effetto distorsivo sulle dinamiche dei prezzi. La Commissione ha altresì preso atto che in numerosi contesti la presenza di asimmetrie informative, la mancanza di trasparenza dei mercati per opacità e incomparabilità dell'offerta (è il caso delle banche e dei diversi servizi finanziari, come risulta dall'audizione della Banca d'Italia e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato), la presenza di reti distributive lunghe costituite da numerosi attori che determinano le variabili di prezzo (è il caso delle filiere alimentari), la costituzione di cartelli più o meno dissimulati, l'inefficienza di organizzazioni distributive onerose ed irrigidite da pratiche che comprimono l'imprenditorialità dei gestori e puniscono i consumatori (è il caso della distribuzione dei carburanti) e, sopratutto, lo scarso affermarsi della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas, e più in generale nei servizi di pubblica utilità, determinano la necessità che Parlamento e Governo assumano le indispensabili iniziative per favorire il migliore dispiegarsi del mercato, le liberalizzazioni necessarie a stimolare la concorrenza e le misure atte a tutelare i contraenti deboli quali i consumatori, soprattutto le fasce più anziane e meno informate della popolazione.

formula alcune conclusioni all'esito di un ciclo di audizioni che hanno avuto ad oggetto problematiche e criticità legate al mercato economico italiano con riguardo alle cause di speculazione che impediscono il libero dispiegarsi della concorrenza e il contenimento dei prezzi delle tariffe, il tutto a scapito dei consumatori finali. Numerosi sono stati gli interlocutori che abbiamo sentito nel corso delle audizioni. I temi trattati sono stati molto vari mi permetto di auspicare per il futuro che la Commissione possa concentrarsi su singoli argomenti da approfondire e studiare con maggior attenzione per ricavare osservazioni e proposte ancora più specifiche. Comunque, dopo due anni di attività della Commissione, possiamo dire che questa maggioranza ha condiviso con noi, in base ai contenuti della relazione conclusiva, la presa di coscienza di un messaggio che arriva chiaro al Parlamento e al Governo. Il nostro Paese ha bisogno di aprire senza indugio la strada ad una nuova stagione di liberalizzazioni per promuovere la concorrenza in mercati che ancora sono chiusi o gestiti in regime di monopolio. Il mercato dei carburanti ne è un esempio calzante. È un settore dominato da otto società verticalmente integrate che, contestualmente, producono, commercializzano all'ingrosso e vendono al dettaglio il prodotto finale: un oligopolio in cui i gestori della rete non sono liberi di approvvigionarsi da altri fornitori a causa del vincolo di esclusiva che li lega alle compagnie petrolifere e, pertanto, non sono in condizione di praticare politiche di prezzo autonome, cosa che non avviene, invece, per le «pompe bianche» di cui si è parlato nel corso delle audizioni, che sono più convenienti e non sono riconducibili ad alcuna compagnia, e si riforniscono sulla base dei prezzi più vantaggiosi. È per questo che, nella conclusione della relazione, il nostro Gruppo ha richiamato la necessità di passare all'esame del disegno di legge n. 2636 - necessità che è stata condivisa quindi anche dalla maggioranza - a prima firma del senatore Bubbico, che formula una precisa proposta legislativa volta ad aumentare la concorrenza nel mercato dei carburanti attraverso la eliminazione dell'esclusiva a carico dei distributori (in tutto o in parte: da vedere sulla base della gradualità con cui applicare questa proposta), cui applicare questa proposta), e attraverso l'assegnazione temporanea all'acquirente unico del compito di esercitare l'attività di commercio all'ingrosso di carburanti per rifornire punti di vendita al dettaglio, che sono appunto liberati dal vincolo di esclusiva. Ogni gestore avrebbe così la possibilità di acquistare combustibili sul libero mercato e praticare prezzi definiti in autonomia. Questa è una delle tante proposte presentate dal nostro Gruppo per la razionalizzazione e la liberalizzazione del mercato dei carburanti. tanto ci sarebbe da fare, soprattutto per superare i vincoli regionali all'accesso alle attività e rendere i gestori veramente imprenditori autonomi da tutti i punti di vista. porterebbero a un significativo contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi a vantaggio del consumatore finale. Altro si potrebbe fare in tal senso: favorire cioè una maggiore trasparenza, garantendo chiarezza e visibilità dei prezzi, rispetto a quanto accade ora. manca, a questo proposito, l'applicazione della disposizione prevista nella legge n. 99 del 2009, in cui veniva conferita al Governo una delega per definire entro sei mesi criteri e modalità per la comunicazione di informazione di prezzo da parte di gestori degli impianti, obbligati appunto a comunicare al Ministero dello sviluppo economico il prezzo praticato per ogni tipologia di carburante. Sarebbe bene che nella relazione conclusiva noi considerassimo ricompreso anche questo auspicio nei confronti del Governo: cosa si aspetta per mettere in atto questa disposizione? Sempre in tema di mercato energetico, la relazione che abbiamo condiviso si sofferma, anche su suggerimento del Gruppo PD, sulla scarsa concorrenza nei settori della produzione e della distribuzione di energia elettrica, ma soprattutto del gas. Da questo punto di vista voglio sottolineare che l'attuale soluzione prospettata dal Governo con l'Atto Senato n. 335 (terzo pacchetto energia) non va nella direzione che è auspicata dal nostro Gruppo parlamentare e sottolineata anche nelle conclusioni della relazione che oggi esaminiamo: il modello di separazione funzionale che è stato scelto dal Governo, infatti, non offre le soluzioni più opportune per lo sviluppo del settore e non garantisce l'effettiva indipendenza tra rete di trasporto e produzione e fornitura. Abbiamo sempre auspicato un modello di separazione analogo a quello del mercato elettrico, e non ci sembra che il Governo stia facendo le scelte competitive per intraprendere questa strada. Vorrei poi sottolineare che, se davvero questa Commissione ha a cuore lo studio dei problemi legati all'aumento dei prezzi nel settore energetico, dovrebbe anche soffermarsi sui problemi legati alle dinamiche inflazionistiche indotte proprio da questo Governo, ad esempio sull'effetto che ha avuto sul prezzo dei carburanti, e di conseguenza anche sull'inflazione - perché abbiamo visto qual è la determinanza dei prezzi energetici sull'inflazione - l'aumento delle accise deciso dal Governo recentemente per finanziare lo spettacolo.

Sempre con riguardo ai temi che questa Commissione ha affrontato e deve continuare ad affrontare, voglio far riferimento ad una precisa formulazione formulazione della relazione. Si legge che i mercati sono caratterizzati dalla presenza di asimmetrie informative, da mancanza di trasparenza, da fenomeni di alterazione della concorrenza e di costruzione di cartelli in grado di alterarla. non possiamo non ricomprendere il settore delle assicurazioni e dei servizi assicurativi, con riferimento alle RC-Auto.

una scarsa mobilità dei clienti tra compagnie e queste possono modificare unilateralmente le condizioni di contratto. Purtroppo, abbiamo visto come al Sud molte compagnie stiano portando avanti una vera e propria politica di disdetta massiva delle polizze, con gravi conseguenze a carico dei contraenti, comunque strozzati da un mercato sempre meno competitivo. Gli automobilisti virtuosi, alla fine, sono i più penalizzati: pagano premi sproporzionati, calcolati sulla base di un parametro territoriale con riferimento al luogo di residenza, per cui assistiamo ad una vera e propria sproporzione dei premi tra il Nord ed il Sud. Qualcosa non funziona, per cui va ripensato il meccanismo *bonus-malus*: dobbiamo conciliare il principio di mutualità con l'universalità della tutela,

Questi sono solo alcuni punti di riforma che riteniamo compresi nella relazione finale e che avete condiviso, dai quali non si può prescindere per dare significato alla funzione e al ruolo della Commissione, che è anche quello di indirizzare il Parlamento e il Governo verso un percorso di riforme che non viene avviato. Non c'è infatti vera attenzione per il tema dei prezzi e per la tutela dei consumatori,

per la sorveglianza dei prezzi, il cosiddetto "mister Prezzi", invece, non ha più alcuna incisività, non esercita la *moral suasion* che ha esercitato nelle legislature precedenti ed è latitante in tutti i casi in cui potrebbe effettivamente intervenire, soprattutto per gli aumenti che riguardano il mercato interno (l'inflazione *core*, come l'abbiamo definita nella relazione). Nelle conclusioni, quando si richiama la necessità di misure atte a tutelare i contraenti deboli e i consumatori, non si può non ricomprendere anche l'attività del Garante dei prezzi. In ultimo, ma non per importanza, come tutti i miei colleghi hanno detto, a ulteriore riprova della scarsa attenzione del Governo sul tema in questione, vediamo qual è il ritardo ormai biennale per l'adozione del disegno di legge annuale sulla concorrenza. Questo Governo si è impegnato a presentarlo nel 2009: ormai ci sembra la solita politica degli annunci e non dei fatti. Allora, che veramente questa relazione arrivi al Governo dal divenire lettera morta, possa stimolare nel più breve tempo possibile l'adozione della legge sulla concorrenza. Signor Presidente, innanzi tutto desidero complimentarmi con la Commissione per l'eccellente lavoro svolto. Mi riferisco in modo particolare all'analisi approfondita ed estremamente corretta

molti sanno che l'agricoltura italiana è la prima agricoltura d'Europa in termini di valore aggiunto, e la seconda d'Europa come produzione lorda vendibile.

i prezzi raggiunti in quel frangente corrispondevano all'incirca ai prezzi che sui mercati nazionali gli agricoltori italiani spuntavano trent'anni prima: prima: di questo stiamo parlando, colleghi. Tutti gli economisti si sono esercitati nel ricercare le cause di quegli aumenti: la speculazione finanziaria, le produzioni bioenergetiche negli Stati Uniti. La conclusione subito dopo le varie analisi, tra la fine del 2008 e i primi del 2009 si è registrato non un decremento sensibile ma un vero e proprio crollo, tra l'altro correttamente riportato nel grafico della Commissione prezzi,

entità del settore alimentare, con particolare riferimento alla fase finale della filiera, specie delle filiere lunghe, tuttora prevalenti nel nostro Paese.

che era cresciuto anche alla luce di quell'aumento assolutamente transitorio del prezzo del grano duro, si è mantenuto alto, nonostante ci sia stato un decremento verticale del prezzo della materia prima. Quindi, la ragione di scambio dei nostri agricoltori è peggiorata in maniera vistosa e il consumatore non ne ha tratto alcun beneficio. Questo, per fatti che hanno riguardato le fasi finali della filiera.

lo ha seguito sia in questo (a volte lo ha anche anticipato), sia nel favorire progetti di filiera corta nonché l'etichettatura del prodotto nazionale, a vantaggio dei consumatori, che almeno potranno scegliere cosa consumare. Questo, per cercare di conservare almeno una parte del valore aggiunto nelle tasche degli agricoltori italiani. Questo è ciò che emerge con assoluta chiarezza dal documento presentato dalla Commissione.

i produttori di pasta a livello nazionale ad un certo punto hanno smesso di acquistare grano duro italiano e si sono rivolti al mercato estero

l'abbiamo voluta noi, il Governo ci ha assecondato e tutte le forze politiche e tutti i Gruppi l'hanno sostenuta. Abbiamo fatto un eccellente lavoro al servizio dell'agricoltura italiana e dei nostri consumatori. Continuiamo così.

senza alcuna polemica con il Presidente, che ha svolto un buon lavoro,

ma, a proposito della famiglia Ligresti e delle tariffe assicurative aumentate del 179,9

i costi di una gestione disastrata, che oggi la banca Unicredit deve contribuire a salvare, e così anche le altre banche.

non ci sarebbe stato il dissesto finanziario che ora bisogna ripianare. Alla fine, a saldare il conto sono stati i poveri piccoli azionisti delle due compagnie. Ricchi premi e *cotillons.* A riempire i portafogli di casa Ligresti negli ultimi anni hanno contribuito i lauti stipendi pagati loro dalle aziende di famiglia. Dal 2005 al 2010 Giulia, Jonella e Gioacchino Ligresti hanno incassato una busta paga complessiva da oltre 60 milioni di euro, 60 milioni di euro, 120 miliardi di vecchie lire, emolumenti pari al triplo della media degli assicuratori europei. Anche l'anno scorso, con i titoli alle corde in Borsa e una voragine da un miliardo nei conti di Fondiaria, i tre moschettieri della famiglia hanno ricevuto una bella gratifica da 8,3 milioni di euro. Ma i compensi sono solo la punta dell'i*ceberg* della pioggia d'oro che hanno incassato direttamente. Fondiaria Sai ha staccato nel 2010 un assegno da 6,7 milioni per consulenze tecnico-amministrative legali a parti correlate. Banca Sai, oltre ad aver finanziato per 19 milioni Sinergia, ha garantito prestiti personali per 3 milioni di euro a singoli amministratori. Qualche spicciolo è finito pure nelle aziende personali dei figli di Salvatore. «Gilli Communication», una società di Giulia, ha fatturato un paio di milioni per le campagne pubblicitarie della Dialogo, una controllata del gruppo Fonsai, mentre Laità, la società proprietaria di Toulon,

gratificata con un pagamento di 1,4 milioni. Questi signori amministratori stanno in 15-20 consigli d'amministrazione. Allora di che parliamo? Parliamo di perdita del potere di acquisto, della CONSOB che non fa il proprio dovere, dell'ISVAP che è disattenta e di un balzo dell'inflazione, che ad aprile è salita del 2,6

su tre milioni di famiglie che hanno contratto mutui a tassi variabili indicizzati, sempre ascoltando i cattivi consigli delle banche. E la Banca d'Italia che faceva? L'ufficio di vigilanza della Banca d'Italia che faceva? Magari commissariava alcune banche, che non obbedivano ai *desiderata* della dottoressa Tarantola, responsabile della vigilanza,

il commissariamento, improvvisamente, finita l'ispezione, si dimette dalla Banca d'Italia e viene assunto dall'avvocato Azzi. Di cosa parliamo in questo Paese?

riguardano i correntisti, i risparmiatori, le imprese che non risorgono neanche nel Nord-Est e alle quali le banche colluse con la Banca d'Italia non danno crediti.

questa Commissione possa andare avanti; però, il Parlamento probabilmente deve fare leggi più stringenti

volevano che fosse venduta ad Abertis. Ce ne circondiamo Presidente? C'è stato qualcuno che si è battuto, anche alcune associazioni dei consumatori: non ne parlo mai, ma anche un Ministro dell'epoca disse che quella operazione non andava fatta e quel ministro si chiamava Antonio Di Pietro.

rappresentante del Governo, come Vice Presidente della Commissione straordinaria controllo prezzi, che si è insediata il 18 dicembre 2008, vorrei ringraziare innanzitutto il presidente Sergio Divina,

a seguito dell'approvazione della mozione a firma dei senatori Bricolo, Finocchiaro, Gasparri ed altri, che ha evidenziato il problema dell'incremento patologico del prezzo dei prodotti petroliferi ed il correlato problema del contrasto del fenomeno inflattivo, temi su cui già il G8 svoltosi ad Osaka nel giugno 2008 si era ampiamente soffermato in relazione agli effetti sull'economia globale. Nello stesso giugno 2008 la Commissione europea ha inoltre invitato gli Stati membri a prendere iniziative a breve termine per sostenere le fasce più povere della popolazione, che risultano essere le più colpite dal fenomeno. L'attività di questa Commissione è oggi ancora più importante, alla luce dell'aumento dell'inflazione rilevato dall'ISTAT. All'insediamento di questa Commissione, l'ISTAT aveva segnato un incremento dell'inflazione, portandola ai massimi livelli dal luglio 1996. Secondo gli ultimi dati, aggiornati ad aprile 2011, l'inflazione continua a correre, mettendo a segno il rialzo maggiore dal novembre del 2008. I beni ed i servizi che hanno registrato maggiori rincari riguardano ancora una volta i prodotti alimentari, i prodotti energetici e quindi tariffe di luce e gas e, con l'avvicinarsi delle vacanze, i trasporti, in particolare traghetti ed aerei. È di questi giorni la notizia riportata da «la Repubblica» che il Garante della concorrenza e del mercato intende verificare il sospetto che le compagnie di navigazione si siano accordate sul rialzo delle tariffe nei collegamenti con la Sardegna, che rispetto all'anno scorso hanno registrato aumenti medi tra il 90 e il 110 Riguardo al rincaro dei trasporti, mi permetto anche di riportare l'esempio dell'aumento vertiginoso del prezzo dei treni. Cito l'esempio di un biglietto di seconda classe Roma-Bolzano, che nell'aprile 2007 ammontava a 47,70 euro e che nell'aprile 2011 ha raggiunto il prezzo di 81 euro, registrando così un aumento del 70 senza alcuna riduzione dei tempi di percorrenza. Chi soffre particolarmente del generale movimento al rialzo dei prezzi dei beni fondamentali sono le famiglie e, in particolare, quelle a reddito fisso che vedono compresso il proprio potere d'acquisto. Gli effetti negativi si riflettono naturalmente anche sul ciclo economico poiché si registra un netto indebolimento della domanda interna. Vorrei sottolineare che anche le associazioni degli agricoltori rimarcano una diminuzione dei consumi che penalizza la redditività e gli investimenti. Ho potuto constatare nelle numerose audizioni che il problema è molto sentito dalle diverse associazioni nazionali, dalle autorità garanti e dalle diverse rappresentanze istituzionali alle quali va il dovuto ringraziamento per il prezioso contributo apportato al lavoro di questa Commissione. Al riguardo, voglio ricordare l'indagine sui beni alimentari nella quale, su richiesta del Garante, la Guardia di finanza ha compiuto accertamenti specifici su alcuni prezzi di vendita di beni o servizi. Sono emersi spesso accordi di cartello fra produttori: ad esempio, al consistente decremento del prezzo del grano sui mercati internazionali non è corrisposta una flessione dei prezzi di farine e semola; di conseguenza, la pasta, come principale prodotto derivato, non ha rilevato nessuna diminuzione del prezzo. L'Autorità garante ha irrogato una sanzione di 12,5 milioni di euro nei confronti degli operatori che hanno concordato politiche commerciali finalizzate all'aumento del prezzo di vendita della pasta secca di semola nel settore distributivo. L'Unione industriali pastai italiani, ascoltata in audizione, ha sottolineato la necessità di considerare tutti i fattori che concorrono alla formazione del prezzo al consumo che riguardano, oltre alla materia prima, anche il costo del lavoro, degli imballaggi, dell'energia, della commercializzazione, del trasporto. Infatti, l'allungamento della filiera, con la presenza di molti intermediari, tende ad incrementare i margini degli intermediatori, producendo consistenti aumenti dei prezzi per il consumatore finale. Al fine di favorire le liberalizzazioni necessarie a stimolare la concorrenza, occorre l'intervento del Parlamento e del Governo. Invito pertanto il Governo a presentare il disegno di legge annuale per il mercato e la

Sud)*. Signor Presidente, illustri colleghi, signor Sottosegretario, voglio ringraziare il presidente Divina e tutti i colleghi della Commissione controllo prezzi, che in questi anni hanno perseguito con costanza lo studio e il monitoraggio dei mercati, approfondendo le dinamiche e le cause relative all'andamento dei prezzi e delle tariffe. È proprio per questo che a nome mio personale e del mio Gruppo dichiaro con convinzione il voto favorevole sulla proposta di

lavoro di analisi su una materia così rilevante quale quella del mantenimento di un corretto andamento dei prezzi nel nostro Paese. Detto questo, in una situazione normale non servirebbe nemmeno una Commissione che vada ad analizzare la concorrenza e l'andamento dei prezzi, perché i prezzi li determina il mercato;

è proprio quella della migliore regolazione dei mercati e, quindi, di una giusta e opportuna concorrenza. Faremo allora alcune considerazioni, sostanzialmente sulle municipalizzate, sui settori della distribuzione e della benzina e sui settori dei servizi.

Il discrimine qui sarebbe molto semplice dal mio punto di vista: una municipalizzata è da tenere pubblica solo se produce utili, ma è da privatizzare subito se genera perdite. E allora si potrebbe richiamare il classico confronto Roma-Milano.

la città di Roma deve invece tappare un buco di 120 milioni di euro, se non di più, causato dalle municipalizzate. Allora, dove bisogna privatizzare? Dove ci sono le perdite, è semplice. il mercato serve per tenere in riga il pubblico, ma non necessariamente il pubblico è da buttar via quando va bene e genera utili. In quest'ottica, è corretta l'impostazione del Governo, che ha previsto la norma che vieta il ripiano delle perdite. Questo, più di tante modifiche normative, andrà a sfoltire l'enorme gruppo di municipalizzate, che altro non sono che carrozzoni e stipendifici pubblici.

di partire alla grande con l'affidamento *in house* di tutti i servizi pubblici, non solo l'acqua. Allora, non si può venire qui a fare i "fenomeni" della concorrenza, e poi andare a dire che è una cosa intelligente fare questa operazione, anche perché se andiamo a vedere i dati - torno sempre alla mia amata Milano - a Milano l'acqua costa meno che in tutta Italia. Negli ultimi sei anni sono stati fatti investimenti che hanno consentito di ristrutturare la rete, ridurre le perdite, e che hanno generato un beneficio per la collettività di un miliardo di euro.

interno dei privati. Questo vuol dire che nell'affrontare un tema spinoso, com'è per esempio quello dei servizi pubblici e come sarà quello dell'acqua, non possiamo comportarci in maniera schizofrenica: qui venire a fare i liberisti e poi in piazza dire l'esatto contrario. altro tema è quello della benzina. È stata affrontata da vari colleghi la questione della liberalizzazione di un mercato che ha una filiera completamente integrata. Vediamo di dare una spinta al disegno di legge a prima firma Sergio Divina, che però ci trova tutti d'accordo, là dove consente al singolo distributore di scegliere da chi comperare la benzina. Questa è una piccola grande liberalizzazione. Mi ricordo quando con il Governo Prodi si fece un'operazione simile nel campo delle assicurazioni. riguardo si poteva porre qualche dubbio, perché l'assicurazione comunque è una componente di servizio, e si poteva eccepire qualcosa. Personalmente sono d'accordo anche sulla completa liberalizzazione di quel servizio.

avvocatura dopo che sono state eliminate le tariffe minime. In quel caso c'è stato un beneficio enorme per i cittadini del nostro Paese dopo l'abolizione delle tariffe minime. Noi Noi qui approviamo all'unanimità una risoluzione in cui si prevede di proseguire su questa strada; però, quando poi si tratta di fare la riforma dell'ordinamento forense, tutti i Gruppi si trovano d'accordo sul reinserimento delle tariffe minime.

Il problema è che però, quando si esce dalle Commissioni e si entra in Aula, prevalgono meccanismi differenti, certe *lobbies* trasversali che alla fine cercano di farla da padrone.

confronto tra le prestazioni delle diverse stazioni di offerta; è necessario un monitoraggio costante sulla formazione di cartelli o di monopoli che alterano il funzionamento del mercato. Non abbiamo problemi di coerenza quando parliamo di liberalizzazione dei mercati. Veniamo da una storia di recenti Governi di centrosinistra che hanno aperto le liberalizzazioni dei mercati. La liberalizzazione dei mercati tutte le volte che si attua produce degli effetti positivi per i consumatori, e in questa relazione mettiamo in evidenza

consumi sotto una certa soglia e per la famiglia media italiana, per le piccole imprese italiane è del 35 per cento più alto di quello dei loro concorrenti europei. Le imprese stanno pagando una situazione di mercato non competitivo, una distorsione del mercato, e lo stanno facendo in termini di mancanza di competitività nei confronti del loro competitori europei. L'andamento e il funzionamento delle banche, secondo l'Autorità di controllo delle banche, cioè la Banca d'Italia, registra spesso un andamento che non va dalla parte del consumatore ma produce volontarie asimmetrie e disuguaglianze informative che colpiscono il consumatore. Noi abbiamo bisogno anche in questo settore di mantenere vigile l'osservazione, così come va, clamorosamente, mantenuta vigile sul settore delle assicurazioni.

Ma è pur vero che siamo di fronte ad un mercato, quello della RC-Auto, obbligatorio per il consumatore, nel quale le assicurazioni (non a mio dire ma a dire dell'Autorità *antitrust*, intervenuta per ben tre volte con delle ammende e sanzioni) hanno un comportamento almeno di cartello rispetto a questo mercato. È vero che vi saranno delle responsabilità anche da parte di fasce di mercato, più alterato nel nostro Paese rispetto ad altri, ma non certamente tale da produrre un 80 per cento in media di costo aggiuntivo della polizza auto in Italia rispetto a quello che avviene negli altri Paesi europei.

prezzi peggiore e più alto rispetto a quello dei servizi tra loro in competizione. Questo vuol dire che le distorsioni organizzative e la posizione di dominanza economica sul singolo mercato locale

Credo che vi sia un problema di coerenza generale nel nostro Paese rispetto alla questione delle liberalizzazioni e dei mercati. È vero che in molte circostanze

Sempre in agguato è il tentativo di bloccare, per consolidare situazioni di dominanza su piccoli e grandi mercati, tanto su quelli professionali, quanto piuttosto su quelli dei prodotti, che dovrebbero essere competitivi. di una difficoltà che dobbiamo superare con determinazione. La Commissione straordinaria controllo prezzi, nelle sue conclusioni, fa un richiamo esplicito al fatto che si vada sempre nella direzione di mettere in moto la concorrenza, perché questa

legato in molte circostanze alla protezione dei propri mercati e delle rendite di posizione. La Commissione controllo prezzi richiama il Parlamento ed il Governo ad affrontare con stabilità e coerenza tutto questo.

e servizi locali, nei quali si sviluppa anche una parte delle cosiddette politiche industriali del nostro Paese. Abbiamo bisogno di mettere in fila tutto ciò, perché il prossimo rapporto della Commissione prezzi agisca magari in totale sintonia con le diverse con le diverse autorità indipendenti che devono agire sui vari mercati: non sono affatto d'accordo sul fatto di mettere le autorità indipendenti nella condizione di essere imputate, di fronte alla necessità che invece abbiamo che siano più forti. In mercati come quelli dell'energia abbiamo

le Autorità intervengano con molta più forza e maggiore determinazione. Un mercato che cresce è competitivo anche perché ha Autorità indipendenti che agiscono per mantenere quella competitività. Evidentemente se cresciamo poco ci saranno responsabilità anche di queste Autorità, ma è certo che minore concorrenza vuol dire minore crescita per il nostro Paese, non solo aumento dei prezzi. Un'inflazione sottile, che passa sui redditi più bassi della popolazione e che li riduce ulteriormente è, come abbiamo detto anche nella discussione di stamattina, una della ragioni della mancanza di crescita del nostro Paese. nostro Paese. Alla fine il cerchio si chiude: mercati più competitivi, Autorità che funzionano nella loro regolamentazione, imprese che effettivamente si misurano con il mercato e con la concorrenza, producono effetti che sono da un lato di trasparenza nel rapporto con il consumatore, di riduzione dei costi e dall'altro effetti di crescita e di implementazione dello sviluppo. In fondo, il messaggio che leggo dalla relazione finale della Commissione è questo: la necessità di un Paese molto più liberalizzato, che a parole tutti vorrebbero ma che nei fatti si persegue pochissimo. Abbiamo bisogno di coerenza. La coerenza va praticata da tutti nello stesso modo, sia a livello locale sia a livello nazionale, che nei confronti degli altri *partner* e degli altri Paesi europei. detto, votiamo a favore di questa proposta di risoluzione, con l'auspicio che il lavoro della Commissione serva da orientamento importante per il resto delle politiche economiche, sulle quali altre Commissioni e il Parlamento tutto devono esprimersi prossimamente e costantemente rispetto all'andamento dell'economia del nostro Paese.

vorrei soffermarmi su una tematica fondamentale nella valutazione della situazione economica del nostro Paese, ovvero il settore energetico, che è anche oggetto delle conclusioni della relazione presentata dalla Commissione.

una particolare valutazione sull'andamento dei prezzi dei carburanti, perché ritengo che riuscire a dominare, anche solo in parte, i prezzi petroliferi, e quindi quelli dei carburanti acquistati dai cittadini, avrebbe un impatto notevolissimo sul bilancio della società, quindi dello Stato. Per meglio comprendere perché il prezzo del petrolio è così volatile, è necessario analizzare una serie di fattori: lo stato delle riserve, il ruolo della geopolitica, l'orientamento dei Paesi produttori, le politiche dei consumatori. Negli ultimi anni si è registrato un forte incremento della domanda di petrolio da parte dei Paesi con limitata capacità produttiva. Se l'offerta è limitata e la domanda aumenta il prezzo del petrolio sale. La scarsa flessibilità del sistema produttivo di affrontare i cambiamenti strutturali per via dell'aumento della domanda porta a sua volta un aumento dei prezzi petroliferi. Ciò che manca nel mercato petrolifero non è il petrolio bensì i suoi prodotti: la capacità di raffinazione nel mondo è limitata a causa dei pochi investimenti in questo settore; il che comporta una carenza di prodotti derivati dal petrolio, soprattutto quelli leggeri come i carburanti, che possono creare tensioni sui prezzi nelle varie aree geografiche. Una delle cause dell'aumento del prezzo del petrolio è il costo della sua lavorazione e non tutte le compagnie vogliono investire in questo senso. Inoltre, la situazione geopolitica, che tende a peggiorare, spinge i produttori petroliferi alla ricerca di nuovi giacimenti in aree più difficili da esplorare, come l'*off* *shore* e le zone di frontiera, e frena gli investimenti nelle aree più promettenti del Medio Oriente, dell'Africa e del Sud America, generando maggiori costi e quindi incrementi del prezzo dei prodotti petroliferi. Altro fattore di influenza sull'andamento del prezzo del petrolio è l'andamento dei cambi e delle borse. Il rapporto euro-dollaro influisce molto sul prezzo del petrolio: aumenta l'euro e diminuisce il prezzo del petrolio e viceversa. Le transazioni che si determinano sulle borse del petrolio non sono solo scambi commerciali (carichi di greggio), ma anche transazioni finanziarie a scopo puramente speculativo senza nessuno scambio fisico. In questo senso le aspettative sui prezzi del petrolio giocano un grosso ruolo e gli speculatori agiscono quando accadono eventi significativi sul mercato, facendo aumentare il prezzo del petrolio e creando distorsioni che modificano l'equilibrio tra domanda e offerta. Il prezzo del petrolio e dei prodotti petroliferi tenderanno a rimanere alti nei prossimi anni, mettendo in difficoltà le economie dei Paesi consumatori che dovranno cercare soluzioni alternative al petrolio per il loro sviluppo economico. Come ben sappiamo, si sta avvicinando il picco di produzione e cioè il momento in cui la produzione di petrolio sarà più bassa della domanda. È già ora possibile sostituire in parte il petrolio con altri combustibili fossili (gas e carbone). I Governi e le compagnie petrolifere guardano più al breve che al lungo termine; per questo mancano robuste politiche di sostegno all'efficienza energetica, alle nuove energie non fossili ed all'innovazione. Siamo arrivati a una svolta di grande cambiamento: i prossimi anni saranno un periodo di transizione dal petrolio verso nuove fonti e tecnologie più efficienti e meno inquinanti, sarà un secolo del grande cambiamento nella sfida energetica mondiale. Le riserve dichiarate, che restano sempre sullo stesso livello, sono in gran parte gonfiate sia dalle compagnie che dai Paesi produttori, per varie ragioni sia di ordine finanziario sia di ordine politico. Sono parecchi anni che le riserve pubblicate indicano sempre in 40 anni la vita residua del petrolio. Per superare questa situazione è necessario ridurre i consumi a parità di servizio reso. Aumentare l'efficienza vuol dire ottenere lo stesso servizio e benessere riducendo i consumi. Il risparmio, ossia spegnere la luce, non dà e non può dare lo stesso benessere. Il prezzo elevato del petrolio è un grande fattore di cambiamento rispetto al passato perché aumenta i costi dell'energia creando squilibri ed inflazione soprattutto nei Paesi più dipendenti e più deboli strutturalmente come il nostro. In tutto ciò bisogna tenere conto anche delle esternalità, ossia le conseguenze dell'uso dell'energia che non ricadono direttamente su chi vende o compra, ma che vanno a gravare su altri attori, in particolare sul pubblico. Per contrastare l'aumento dei prezzi occorrono politiche forti sull'offerta e soprattutto sulla domanda, accordi tra Paesi produttori e consumatori, una revisione della forte fiscalità su quasi tutti i prodotti e, soprattutto, la ricerca di base e tecnologica per trovare nuove fonti di energia a basso costo. Per questo la Commissione straordinaria per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati ha svolto un lavoro molto interessante ed attento per meglio definire la politica nazionale, per contrastare l'inflazione e l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dei carburanti (che si ripercuotono particolarmente sulle famiglie) e per migliorare, quindi, la disciplina in materia di sorveglianza dei prezzi praticati ai consumatori finali. Ricordo che in Italia l'inflazione ha registrato in questi ultimi anni una accelerazione provocata in prevalenza dalle componenti alimentari ed energetiche, che incidono sull'indice generale dei prezzi al consumo per una percentuale pari al 25 per cento. In particolar modo, nel secondo semestre del 2010 le dinamiche inflazionistiche sono state influenzate dalle componenti energetiche e dalle oscillazioni del valore del petrolio greggio sui mercati internazionali. Concordiamo quindi con quanto asserito nelle conclusioni della relazione, nel punto in cui afferma

favorendo l'imprenditorialità, la concorrenza e la tutela dei cittadini che, non dimentichiamolo, sono spesso disorientati da variazioni a volte giornaliere dei prezzi di alcuni beni come la benzina da autotrazione. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo PdL, ringraziando ancora una volta la Commissione per il lavoro svolto, nella certezza che il Governo, come sempre, agirà fattivamente nell'ottica del benessere comune. Onorevoli colleghi, vi informo che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti del Liceo classico «Francesco Vivona» di Roma, ai quali diamo il benvenuto.

sulla comunicazione congiunta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo: "Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale"***

nascono dal particolare momento nel quale questa stessa risoluzione è stata adottata e soprattutto dall'esigenza di di consentire la partecipazione di un ramo del Parlamento, in questo caso del Senato, al processo di definizione di una decisione europea promossa dalla Commissione, che si sviluppa secondo le nuove modalità del Trattato di Lisbona anche - come è a tutti noto - attraverso il ruolo e la funzione dei Parlamenti nazionali. Le ragioni di intervento tempestivo derivano dal fatto che la risoluzione si esprime su un'iniziativa della Commissione relativa ai fatti che hanno caratterizzato la storia dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo nei mesi più recenti. Come noto, il cosiddetto risveglio dei popoli della sponda Sud del Mediterraneo presenta differenze; è stato in vario modo spiegato, ma comunque ha un punto fondamentale ormai inequivocabile: nessuno lo aveva previsto in questa forma e con queste modalità. Per tali ragioni, la Commissione, nell'ambito dell'Unione europea ha tempestivamente promosso una sua proposta, che ha chiamato con un nome molto impegnativo: una comunicazione per costruire - cito testualmente «Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale». Il titolo, come già evidenziato, è impegnativo, ma contiene contiene in sé un'intenzione ed uno sforzo sicuramente encomiabili e da condividere. Nell'esame più preciso dei contenuti della proposta della Commissione europea, all'interno della 3a Commissione e d'accordo con il Governo, abbiamo rilevato alcuni elementi, che adesso ripropongo all'attenzione dell'Assemblea, che noi giudichiamo importanti, sia negli aspetti di condivisione, ma anche in quelli di critica. critica. Tutto ciò va inquadrato in un contesto nel quale le novità intervenute in ambito regionale sono assolutamente importanti, così come la tempestività che ha mosso la Commissione a dare questa comunicazione. Il primo punto da sottolineare è che abbiamo condiviso positivamente l'iniziativa della Commissione.

e soprattutto la consapevolezza che il cosiddetto risveglio - come viene definito - è basato su presupposti che trovano una loro ragione in questioni di natura economica, sociale, di libertà e di democrazia. Da questo punto di vista emerge un primo elemento di cambiamento importante, che riteniamo debba intervenire nell'azione dell'Unione. Occorre abbandonare la pretesa di ieri

Questa linea politica si è rivelata del tutto errata e per niente adeguata a ciò che in quei Paesi stava maturando. Questo, quindi, è un primo elemento di cambiamento.

Non c'è l'obbligo della presenza. Prima di tutto l'inquadramento strategico di questa posizione. Questa comunicazione è inquadrata all'interno della politica di vicinato che, come sappiamo, è una delle politiche che l'Unione europea ha nel suo *carnet* di iniziative. La nostra valutazione è che la politica di vicinato rivolta ai Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, per tutto quello che sta succedendo e che potrà succedere, non è adeguata, è una politica debole.

una politica di partenariato per la democrazia e soprattutto per la prosperità, perché per produrre la prosperità - lo dice la parola stessa - è necessario non avere solo buone intenzioni, ma anche risorse adeguate.

tra le priorità nelle iniziative dell'Unione e che al contrario, alla luce di quanto sta accadendo, dovrebbero essere rilanciate. Inoltre, di tutti i nuovi strumenti previsti dal Trattato di Lisbona alcuni sono stati impiegati in maniera in maniera inappropriata, mentre altri non sono stati per nulla applicati nella nuova situazione che si è determinata. Valga per tutti, ad esempio, come l'Unione si è mossa nell'affrontare il tema dell'emergenza emigrazione. L'ultima comunicazione della Commissione del 4 maggio in risposta ad una sollecitazione venuta da singoli Paesi e anche dal documento congiunto Italia e Francia, che è prodotto a seguito del recente *summit* che si è svolto in Italia nel mese di aprile, esprime ancora una volta l'inadeguatezza delle modalità con le quali la Commissione approccia questo problema così come si sta delineando e così come si è delineato finora, per cui, in assenza di cambiamenti profondi, si rischia di produrre ulteriori elementi negativi in futuro. Non è mettendo in discussione gli accordi di Schengen, o lasciando che i singoli Paesi mettano in discussione Schengen che questa questione può essere affrontata; né tantomeno possiamo immaginare che una generica politica di solidarietà alla quale ci richiamiamo in casi come questi possa essere la medicina che risolve il problema. ci sono nell'ambito dei trattati degli istituti che possono essere impiegati e rilanciati, e noi pensiamo che da questo punto di vista la risoluzione proponga alla Commissione una riflessione più approfondita su questi temi, che la rende capace di uscire dall'ambito di inadeguatezza che finora si è determinato. che integrano la relazione scritta, servono a mettere in evidenza che noi pensiamo di offrire al Governo, in vista del prossimo Consiglio del 24 giugno, una valutazione in sede parlamentare che rafforzi l'iniziativa che il Governo italiano ha finora profuso in questa direzione (in particolare, per tutto ciò che ha riguardato l'emergenza immigrazione che ha visto l'Italia assolutamente in prima linea), consapevoli del fatto che esiste un'insufficienza nell'azione svolta anche dall'Alto rappresentante, nuovo istituto introdotto dal Trattato, in tutta la vicenda così com'è si è sviluppata finora, sia nelle sue iniziative politiche che nei documenti che ha proposto. Da questo punto di vista occorre che, poiché l'Alto rappresentante è anche il Vice Presidente della Commissione, si registri un cambiamento d'atteggiamento volto a fornire una risposta coordinata a livello europeo di tutte le politiche che sono necessarie in questa direzione. La situazione nel Mediterraneo nel complesso, quindi, impone una politica estera e di sicurezza più coordinata ed efficace, che sappia utilizzare appieno i nuovi strumenti previsti dai trattati, in questa prospettiva, secondo la Commissione esteri, occorre, a fianco del processo negoziale relativo all'adesione in quel quadro di cambiamento e rilancio della politica multilaterale, venga coinvolta in modo attivo nella definizione di questo pezzo di politica estera dell'Unione. Queste sono le motivazioni generali che, aggiunte a quelle contenute nella relazione, hanno ispirato la risoluzione che la Commissione esteri

negli anni Sessanta e Settanta. Si continua cioè a parlare di diritti dell'uomo. Diciamo che oggi possiamo permetterci la traduzione letterale dall'inglese, se non vogliamo affrontare la questione dal punto di vista culturale, e parlare di diritti umani proprio perché appartengono anche alla donna. Se vogliamo promuovere delle strategie che abbiano a che fare tanto con la promozione della democrazia quanto con la prosperità e non garantiamo diritti e libertà alle donne, cioè alla metà alla metà di qualsiasi area geografica di cui si voglia parlare e in particolare in Medio Oriente e in tutta l'area del Mediterraneo, sicuramente né democrazia né prosperità possono essere considerate obiettivi raggiungibili. Dico questo proprio in virtù delle ultime sommosse che hanno caratterizzato quella che viene ormai classificata su tutti i giornali una "primavera" mediorientale o araba, perché non di rado si ritiene che uno dei motivi per cui tutto ciò è nato sia da ravvisare nella mancanza di di *status* sociale ed economico di buona parte di coloro i quali sono scesi in piazza per protestare contro i regimi autoritari e dittatoriali che vigevano in Tunisia, in Egitto, in Libia, in Siria, in Yemen, in Bahrein molto probabilmente nelle prossime settimane continueremo a vedere questo tipo di sommovimenti ampliarsi fino ad arrivare, che so, in Mauritania, in Ciad e, speriamo, un giorno uscire dal mondo arabo e arrivare anche in Iran). La povertà è spesso frutto di vari fattori. Sicuramente ci sono problemi inerenti all'economia, che nei Paesi del Nord Africa è sfavorita, non soltanto da condizioni geografiche, ambientali e climatiche particolarmente poco indicate per coltivare in maniera intensiva ed estensiva tutta una serie di beni; ma la povertà oltre che di un altro problema che toccherò più avanti, di una vera e propria esplosione demografica che negli ultimi trent'anni ha caratterizzato quella regione, facendone un luogo ultrapopolato e, in virtù della povertà e della finta promessa di un lavoro in zone urbane, ad altissimo tasso di urbanizzazione progressiva. Tale urbanizzazione da un lato ha creato megalopoli invivibili, ingovernabili totalmente mancanti di qualsiasi tipo di struttura, dall'altro ha desertificato quelle parti di terra che avrebbero potuto essere coltivate e quindi avrebbero potuto contribuire al sostentamento o alla creazione di economie - per lo meno per quanto riguarda l'agricoltura - autosufficienti in buona parte di questi Paesi. Se mettiamo insieme, appunto, da una parte i problemi economici e, dall'altra, l'esplosione demografica che ha caratterizzato questi Paesi, e li includiamo nella totale mancanza di rispetto dei diritti fondamentali, di certezza del diritto e quindi di pratica democratica quotidiana, ecco che abbiamo un contesto in cui occorre avviare una lettura che includa questo problema nella ricerca di soluzioni possibili, ma altrettanto sicuramente fare sforzi ben superiori rispetto a quelli che

La Commissione ha elaborato un documento che non soltanto tiene conto di quanto è stato detto dal Consiglio e dalla Commissione ed è successo nel mondo, ma, credo, ha anche dovuto tenere conto delle azioni e delle iniziative che questo Governo ha ha cercato di portare avanti nei mesi scorsi per far fronte a un contesto che in molti ritengono ancora oggi - ahinoi - essere una sorpresa, mentre chi segue con meno disattenzione le questioni mediorientali si è da sempre posto come una delle possibilità Il Governo italiano credo continui - e questo gli è stato sempre riconosciuto da tutti, maggioranza, minoranza, opposizione e opposizione dell'opposizione, come per esempio chi vi parla - a mantenere, se non altro a parole, una grande attenzione al *partner* strategico più importante dell'area euromediterranea, ricordato anche dal senatore Cabras, e cioè la Turchia.

soluzioni di crisi che invece che perpetuare la stabilità che ha portato la sottomissione, spesso anche *manu militari*, di centinaia di milioni di persone (una stabilità fondata sulla ricerca del bilanciamento, se non altro nel breve-medio periodo, di un contesto che non ha mai conosciuto libertà) favoriscano l'evoluzione di un contesto che invece inizia ad assoggettare gli individui alla legge, piuttosto che ai carri armati (come invece continuiamo a vedere in queste ore in Libia, e credo ancor di più in Siria). La Turchia quindi - e lo dice espressamente il Documento - deve essere coinvolta dai 27 Stati membri dell'Unione europea ogniqualvolta si prendano decisioni relativamente alle direttive di maggiore importanza in tema di politica estera comunitaria; ma è una Turchia che deve essere coinvolta tanto all'interno della Unione europea quanto all'interno della NATO e quanto, altrettanto sicuramente, all'interno del lavoro che occorre le democrazie riprendano in seno alle Nazioni Unite ogniqualvolta si parla di diritti umani, di promozione della democrazia e, ancor di più, di promozione della prosperità.

ancora, fortunatamente, prevalentemente laico, può essere uno dei migliori *partner* nella ricerca di dialogo anche a livello religioso. Il Governo italiano, però, non credo possa essere portato ad esempio di comportamento relativamente alla prevenzione o gestione di altri tipi di emergenze che si sono verificate negli ultimi due mesi, non soltanto perché all'indomani della prima rivolta di piazza tunisina il ministro Frattini ebbe modo di dire che il modello che dovrebbe valere per il Nord Africa era quello della Libia, cioè di un controllo della popolazione, non soltanto quella nazionale ma soprattutto quella non nazionale, che avrebbe potuto avviare una serie di flussi migratori verso il Nord, ma perché, tanto con il regime di Ben Ali quanto con il regime di Mubarak, l'Italia ha sempre mantenuto un rapporto di equilibrato vicinato per alcune questioni ma, molto probabilmente, di altrettanto coraggioso (detto col senno di poi) sostegno di alcuni tipi di politiche, tanto che l'Italia era andata a finanziare una scuola di giornalismo a Tunisi, in un Paese in cui esisteva la censura e dove venivano messi in carcere *blogger* nei giorni in cui le Nazioni Unite, nel 2005, organizzavano il *summit* mondiale sull'informazione. Si tratta di persone che, una volta in carcere, solo grazie alla partecipazione di molte ONG internazionali, ad una parte della società civile tunisina che non voleva sottomettersi alla politica di Ben Ali e grazie anche alla non violenza - vi furono scioperi della fame di giorni e giorni - sono riuscite a far conoscere, alla fine, qual era la vera realtà nel campo della libertà d'informazione tunisina. Purtroppo, l'Italia ha continuato a finanziare quella scuola di giornalismo, in un Paese in cui non si poteva dire quel che si voleva perché altrimenti Ben Ali e la sua famiglia si sarebbero sentiti offesi e avrebbero reagito mettendo in carcere chi cercava di promuovere tutto quello che poi, invece, da tre settimane, l'Italia *in primis* ma anche gli altri Paesi europei ritengono essere il futuro necessario per la Tunisia. L'ultima questione che volevo affrontare, visto che il tempo a mia disposizione è finito,

una grande iniziativa, sicuramente italiana (non solo perché siamo i più vicini all'Africa) ma altrettanto sicuramente, come minimo, di tutti i Paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo. Infatti, ancora oggi si sentono falsificare i dati, si sentono manipolare le poche informazioni reali circa la qualità di chi fugge, e si lascia alla propaganda, piuttosto che alla certezza normativa, il governo di questo fenomeno, che credo nei prossimi mesi possa diventare ancora più grave, e non fosse soltanto per il fatto che si va incontro alla bella stagione e, quindi, le condizioni del mare consentiranno maggiori sbarchi.

*(PD)*. Signora Presidente, interverrò solo su alcuni aspetti fra quelli trattati nella relazione dal senatore Cabras.

Non possiamo dimenticare che almeno dalla fine degli anni '70, ossia da quando il presidente Sadat ha concluso l'accordo di pace con Israele, la grande coalizione fra Occidente e arabi moderati è stata uno dei pilastri delle politiche di sicurezza che hanno orientato il nostro mondo. Oggi tutto questo non è più certo. Oggi tutta la questione è completamente aperta.

coincideva con la difesa di quei regimi, anche con tutte le loro brutture, e non rifarò gli esempi già fatti.

dell'Islam fondamentalmente attraverso le lenti della lotta contro il terrorismo e il fondamentalismo. Attraverso queste lenti non siamo riusciti a comprendere quanto stava cambiando in quelle società. Stava cambiando qualcosa di profondo.

delle forze che l'hanno messa in moto, forze nelle quali l'ispirazione democratica e la battaglia per la libertà sono state il tratto caratteristico. che questo processo si è sviluppato - naturalmente l'analisi dovrebbe riguardare i diversi Paesi - la situazione è diventata più complessa. Sono entrate in campo forze più strutturate e naturalmente alla spinta per la democrazia e la libertà si sono aggiunti molti fattori.

nel determinare cioè se questo movimento fondamentale si dirigerà verso la libertà, la democrazia e manterrà le promesse

vede oggi una drammatica crisi della politica europea: in un momento in cui ci sarebbe un'esigenza così importante e così forte di un intervento politico dell'Europa, siamo di fronte ad un'Europa che politicamente non esiste, ad un'Europa che va in ordine sparso ai diversi appuntamenti e che non riesce a esprimere una politica comune. Questo mi pare il punto più significativo. Scegliere di svolgere questo ruolo politico comporta alcune scelte di fondo. di rimettere in discussione quella pretesa di *realpolitik* che si è dimostrata molto poco realistica. Lo dico al sottosegretario Scotti: oggi c'è un punto su cui alle parole bisogna mostrare di far seguire qualche fatto, questo punto si chiama Siria.

di una politica più forte e che consideriamo questi fronti come strategici e poi, nelle scelte concrete che facciamo, tagliare ogni volta in modo drammatico le risorse a disposizione delle politiche in questo campo. Naturalmente ci sono le politiche multilaterali, ma ogni Paese ha bisogno di coltivare, attraverso le proprie iniziative bilaterali, una politica in questa direzione. Non lo stiamo facendo abbastanza, e questa può diventare non solo un'occasione persa per ogni Paese ma anche una responsabilità molto pesante rispetto alle possibilità di ricostruire una nuova dimensione della sicurezza. Sappiamo che stiamo facendo questa discussione in un momento in cui tante variabili sono completamente in movimento.

a forze palestinesi unite di aprire sul serio una trattativa di pace con Israele, o andrà nella direzione contraria? Sono tutte questioni aperte, su cui ci vorrebbe un'iniziativa politica più forte alla quale oggi stiamo assistendo. Penso che la discussione che stiamo facendo abbia questo senso: quello di spendere il peso e l'influenza del Senato e del Parlamento italiano

*(IdV)*. Signora Presidente, volevo portare all'attenzione dell'Aula e anche dell'opinione pubblica, che ascolta i nostri lavori tramite Radio Radicale, la questione di "Iniquitalia" (altro che Equitalia, bisogna chiamarla "Iniquitalia"), oggetto di proteste e manifestazioni di piazza per i metodi di riscossione dei tributi che rasentano l'estorsione (ripeto, la vera e propria estorsione). Ogni giorno leggiamo sui giornali di proteste. A Cagliari, in Sardegna, decine di migliaia di lavoratori hanno protestato

una moratoria; il sindaco Emiliano di Bari addirittura non intende più fruire di questi servizi di veri e propri estortori. Cosa succede? Questi non vanno tanto per il sottile, mettono ganasce fiscali al di sotto di quanto non abbia stabilito una recente sentenza di Cassazione per tributi come qualche contravvenzione di 70, 80 o 100 euro, che è oneroso contestare perché bisogna rivolgersi per esempio ad un numero a pagamento che non risponde mai oppure bisogna recarsi in quel girone infernale delle agenzie. Invito i senatori ad andarci,

imposto spesso riscossioni che non dovrebbero esserci. Questa montagna di multe, 14 milioni, sta piegando le spalle dei cittadini. Sono un milione Sono un milione e mezzo ormai gli immobili con un'ipoteca giudiziale iscritta al registro immobiliare; 426.000 le ipoteche degli ultimi tre anni. Si tratta di artigiani, commercianti, gente onesta, non dei grandi evasori (quelli con i quali Equitalia e le Agenzie delle entrate si genuflettono, che portano i capitali all'estero): è la povera gente! Quindi ho presentato, anche con il mio Gruppo, un disegno di legge per istituire una Commissione d'inchiesta e ho presentato numerose interrogazioni parlamentari. Mi auguro che questo Governo, che fa il Robin Hood alla rovescia, venga a rispondere e possa mettere fine, sanzionandoli, anche a questi comportamenti. Signora Presidente, attenzione, andate negli uffici. Non è colpa degli impiegati (il direttore Befera ha detto che sarebbe colpa degli impiegati): questi si prodigano per risolvere le questioni! È colpa delle direttive e di un sistema fiscale

All'indomani dei risultati elettorali, il Presidente del Senato ha ritenuto utile e opportuno non commentare ciò che era uscito dalle urne. Purtroppo però lo stesso atteggiamento da tre mesi e mezzo viene tenuto dal Presidente del Senato relativamente alle richieste di notizie circa il bilancio interno della nostra Camera. è il 18 maggio. Io vorrei sapere, anche perché un mese fa era stato detto che il Collegio dei senatori Questori aveva licenziato il documento, che fine abbia fatto il passaggio al Consiglio di Presidenza.